La seduta è ripresa. La seduta è ripresa.

apre una nuova finestra"). L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Signora Presidente, vorrei innanzitutto omaggiare le popolazioni indigene, aborigene, native degli Stati Uniti, che giustamente rivendicano un'attenzione particolare nei loro confronti per quello che storicamente,

il significato dei sacrifici ed esaltando comunque l'apporto delle comunità che fanno parte integrante oggi degli Stati Uniti,

delle comunità aborigene, sia nei confronti della popolazione che venne strappata all'Africa, sia nei confronti degli italiani, sono durati per secoli e hanno coinvolto grandi personaggi, come Jefferson, Washington, Lincoln,

intessuta di ignoranza dei fatti storici e di ideologia, che vuole cancellare il contesto storico in cui determinati avvenimenti si sono svolti, con una furia iconoclasta che assomiglia a quella dell'ISIS e dei talebani quando vanno a distruggere

veramente singolare, che fa pensare fin dove ci si voglia spingere attraverso questa *damnatio memoriae* di tutto quello che è stato il passato.

ai milioni e milioni di persone che hanno contributo a costituire l'America di origine italoamericana e - soprattutto - è a fianco a coloro che fanno una battaglia di verità su questo delicato argomento.

prima di inoltrarmi nell'argomento oggetto della discussione, mi consenta, ancora una volta, di rivolgermi alla sua cortesia per segnalarle che l'impianto microfonico che divido con il collega nel mio seggio

A pochi giorni dalla rievocazione della data in cui Cristoforo Colombo sbarcò in America - il 12 ottobre 1492 - ci sentiamo di condividere il contenuto

come gli Stati Uniti d'America, hanno un valore simbolico e possono muoversi solo attraverso i canali della diplomazia. Ecco, però, Ecco, però, che il dibattito odierno - assieme alla condanna unanime delle persone di buon senso di ogni forma di violenza - può essere un utile strumento per contrastare ed emarginare l'ignoranza di chi vuole eliminare i simboli del passato. La storia non si cancella e soprattutto non si riscrive, in assenza di ricerche e approfondimenti ponderati e ben documentati. Rileggere ora, dopo cinque secoli, la vicenda, le azioni e il pensiero di Cristoforo Colombo, con un approfondimento da *social network* (una volta si sarebbe detto da bar dello sport) è un atteggiamento che lascia molto perplessi. Non possiamo però non rilevare che questa superficialità e questa faciloneria hanno comportato danneggiamenti concreti a luoghi e simboli della storia americana. americana. Alla irresponsabilità bisogna rispondere con la cultura della ricostruzione storica e con la consapevolezza dei fatti. La tradizione storica attribuisce al mio concittadino genovese Cristoforo Colombo la scoperta dell'America. In realtà, sappiamo benissimo che le Americhe erano abitate da secoli e che quando Colombo e i suoi uomini sbarcarono sulle coste delle odierne Bahamas trovarono delle popolazioni indigene con cui dovettero confrontarsi. Se le navi spagnole, guidate da un grande genovese, non fossero giunte sulle coste americane alla fine del Quattrocento, ci sarebbero arrivate altre spedizioni qualche anno dopo, come effettivamente fu, e il confronto-scontro con le popolazioni indigene - che va letto con gli strumenti culturali di quei tempi, non con quelli di oggi - sarebbe stato lo stesso che ebbero con loro Colombo e i suoi marinai spagnoli. Del resto, il grande genovese fu incarcerato e processato per le presunte violenze o uccisioni di nativi americani. Fu prosciolto e giudicato innocente dai giudici e con i codici del suo tempo. Non ha quindi alcun senso celebrare processi sommari, lontani cinquecento anni dai fatti e con i codici di oggi, come qualcuno demagogicamente vorrebbe fare. Egli non morì ricco e non trasse grandi guadagni in danno di qualcuno dalle sue navigazioni, cosa che per un genovese è quantomeno anomala, né dalla scoperta che ha cambiato il mondo. È stato celebrato principalmente perché si ritenne importantissimo il suo contributo alla colonizzazione - termine che oggi viene letto dai più come evidentemente non positivo Quegli americani che ora protestano contro i simboli legati alla scoperta e alla conquista della propria terra da parte dei primi pionieri europei, finiscono col calpestare la propria stessa storia, che è quella di un grande popolo laborioso, fatto di coraggiosi pionieri e inventori, proprio come Colombo. Diverse città americane stanno tuttavia cancellando i festeggiamenti del Columbus day, per prevenire ed evitare possibili scontri e violenze da parte di frange oltranziste. Festeggiarlo oggi, però, significherebbe celebrare il sogno di ogni americano - dalla rivelazione del nuovo mondo alla invenzione dell'algoritmo di Google - che può realizzarsi in una Nazione straordinaria, da cinquecento anni, anche grazie alla scoperta di Cristoforo Colombo.

ma un'eredità culturale dell'umanità, essendo un pioniere del mondo nuovo. Va riaffermata la figura di un grande uomo, emblema della navigazione e delle scoperte scientifiche. Cristoforo Colombo è, inoltre, per la comunità italiana e italo-americana un simbolo di coraggio e intraprendenza, che abbiamo il dovere di difendere e sostenere. Lo dobbiamo alle generazioni di emigranti italo-americani, arrivati in America dopo Cristoforo Colombo e a quelle che verranno in futuro.

ha detto: «L'esploratore è un Ulisse moderno, è il simbolo della nostra forza di volontà, di iniziativa individuale e della curiosità per il nuovo. Valori universali che hanno da sempre reso orgogliosa la comunità italiana e che hanno contribuito a costruire il nostro sogno americano affrontando con essi i momenti più difficili». Le posizioni critiche sulla figura di Cristoforo Colombo hanno raggiunto un livello inaccettabile, producendo iniziative iconoclaste che, inizialmente rivolte contro le statue dei generali sudisti e schiavisti sconfitti nella guerra civile, hanno preso di mira statue e raffigurazioni. casi sono stati citati e non li ripeto. Va riconosciuto comunque che il presidente Trump, proprio nel programmare la celebrazione del Columbus day, ha voluto esprimere un forte sostegno alla figura

Noi riteniamo la figura di Cristoforo Colombo significativa nella storia americana, in quanto, al contrario della visione di chi sostiene la protesta, ha dato un forte e positivo contributo alla maturazione della democrazia, alla lotta contro ogni forma di discriminazione e all'integrazione culturale e sociale, attraverso le rappresentanze dei popoli europei presenti sul territorio americano. Quindi noi con questa mozione chiediamo che, mediante le proprie rappresentanze consolari, la comunità italoamericana sia supportata nella sua protesta e che, per il legame di amicizia che ha sempre contraddistinto il dialogo tra l'Italia e gli Stati Uniti, venga data una corretta lettura del significato e del valore che figure storiche come Cristoforo Colombo portano con sé. Questo sostegno si determina soprattutto mediante iniziative, in collaborazione con le comunità italoamericane, con i centri studi e con le università, tese ad approfondire una figura che merita, attraverso la conoscenza storica, la massima integrità e l'assoluta dignità della memoria.

onorevoli colleghi senatori, da cittadina ligure e da cittadina italiana non posso che sottoscrivere con convinzione una mozione che impegna il Governo, attraverso la sua rete diplomatica consolare, a valorizzare e sostenere negli Stati Uniti la figura del grande esploratore Cristoforo Colombo. Come noto, i recenti episodi di intolleranza verso alcuni simboli della storia americana e il conseguente dibattito accesosi nella società, che in Italia è giunto sulle pagine dei giornali, hanno colpito anche diverse statue raffiguranti il celebre navigatore genovese, che negli Stati Uniti è considerato un'icona da parte degli italoamericani, che ne festeggiano la memoria il secondo lunedì di ottobre. A Baltimora, a Detroit, a Houston e in altre città minori si sono registrate azioni dimostrative, mentre a Los Angeles il consiglio comunale ha votato a favore di una mozione per la cancellazione del Columbus day e perfino a New York si sta discutendo

quando la Compagnia di St. Tammany organizzò una serie di festeggiamenti per commemorare il 300° anniversario della scoperta dell'America. La stessa festa venne ripetuta nel 1892, riconosciuta nel 1937 dal presidente Roosevelt e infine, nel 1971, dichiarata festa nazionale dal presidente Richard Nixon, da celebrarsi con parate e festeggiamenti

Lo stesso ex presidente Obama, nel 2012, in occasione del suo discorso per le celebrazioni del Columbus Day, sottolineò come Cristoforo Colombo sia stato un esempio che ha ispirato generazioni di immigrati italiani, spingendoli a seguire le sue orme, per poi celebrare gli innumerevoli contributi che tante generazioni di italoamericani hanno dato alla Nazione americana. E Cristoforo Colombo è anche un simbolo per parte della comunità ispanica, che rivendica un infondato Colombo spagnolo e il contributo della Corona di Spagna alla scoperta del continente americano. La più recente storiografia su Cristoforo Colombo - questo va detto - ne fa emergere una personalità discutibile, macchiatosi di comportamenti violenti e crudeli nel rapporto con gli indigeni delle terre da lui scoperte. Un'immagine, quindi, ben diversa dall'iconografia classica che tutti noi abbiamo studiato sui libri di scuola. Anche la tratta degli schiavi, secondo alcuni storici, fu avviata proprio da lui. Questo ha portato, negli ultimi anni, a considerare anch'egli un simbolo dell'oppressione nei confronti delle popolazioni native e del loro sterminio. Tuttavia mi sembra palese che operazioni come queste, e mi riferisco alla rimozioni di simboli e di statue, non abbiano alcun senso. Quello che la nostra diplomazia dovrà fare, negli Stati Uniti, è adoperarsi affinché si possa rileggere la figura di Colombo con il necessario equilibrio, nei libri e nei programmi scolastici,

tra l'Italia e gli USA, una relazione viva e vibrante che tutti noi vogliamo preservare e portare avanti. Nessuno nega gli orrori dei *conquistadores* e la tragedia che ha colpito le popolazione native e indigene, ma cancellare Cristoforo Colombo, in ossequio al politicamente corretto, è francamente ridicolo.

a intervenire per fare una notazione. Non conosco l'albero genealogico di de Blasio, attuale sindaco di New York, ma il nome non ha bisogno di ricerche araldiche particolari per ascriverlo,

avendo le conoscenze e le qualità, può scrivere libri e fare conferenze), ma addirittura l'architettura del nostro Paese, distruggendo simboli e monumenti che non hanno una valenza ideologica ma sono la testimonianza di un'epoca. Io, però, voglio dare atto del fatto che, mentre l'originario italiano de Blasio, sindaco di New York, ha partecipato a questa campagna di contestazione di simboli e statue che vedono in Cristoforo Colombo, per varie ragioni che non è necessario sottolineare, il simbolo principale, il presidente Trump (del quale pure non conosco l'araldica e le origini, ma certamente Trump non ha origini italiane e questo è abbastanza evidente) ha detto in questi giorni: «Nel Columbus day noi onoriamo l'esperto navigatore e uomo di fede, la cui coraggiosa impresa ha unito due Continenti e ha ispirato molti altri, contro ogni dubbio o avversità». Il presidente Trump generosamente rinnovato e ribadito le espressioni di amicizia tra gli Stati Uniti d'America e l'Italia, testimoniate anche da questi vincoli, etnico-storici che sono di natura originaria, perché Cristoforo Colombo, navigando forse

a quelle di New York). C'è anche Colombo, per fortuna, e quindi Trump, nonostante le visite, francamente più folcloristiche che di valore che Renzi ha organizzato, portandosi dietro la Nicolini Benigni, ha trovato questi motivi. Vorrei anche dire a quelli che fanno battaglie sul passato in Italia e in America che poi dovrebbero cambiare anche il nome al continente americano, perché qui si parla di Colombo, ma l'America - qui c'è l'illustre vice ministro Giro che è impegnato in varie battaglie, ma lo vedo in buona salute nonostante la dedizione con cui si dedica a cause sulle quali abbiamo opinioni diverse, ma nel rispetto reciproco da Amerigo Vespucci, altro noto navigatore che circumnavigò il Continente americano. Da lì è venuto il nome dell'America, così come il Venezuela prende il nome da Venezia e potrei citare molti altri esempi.

i più importanti dei quali poi aprirono la strada alle moderne telecomunicazioni, quelle che ci consentiranno, forse, attraverso qualche *social network* o altri canali, di dire a de Blasio: scendi sul pianeta terra, ricordati dei tuoi antenati e rendi omaggio all'Italia e a Cristoforo Colombo.

Il Columbus day ha consolidato negli anni il carattere di celebrazione dedicata alla collettività italoamericana negli Stati Uniti e al suo contributo nello sviluppo del Paese. Esso si celebra con importanti manifestazioni, quali parate, cortei e discorsi pubblici, in grandi città come New York, San Francisco e Chicago, e vasta partecipazione popolare da parte di italoamericani e sostenitori dell'*italian way of life* d'Oltreoceano. Cristoforo Colombo è diventato, quindi, il primo, storico simbolo della progressiva integrazione e affermazione, dapprima dei nostri emigrati e, con il passare delle generazioni, di una comunità italiana sempre più presente anche a livelli apicali nella società, nella politica, nell'economia e nella cultura degli Stati Uniti d'America. Negli Stati Uniti è in corso da alcuni anni un dibattito, alimentato da ambienti legati ai nativi americani, che mira all'abolizione del Columbus day, per sostituirlo con Giornate delle popolazioni native, alla luce di una rilettura della storia americana successiva al 1492, secondo la quale la spedizione di Colombo avrebbe assoggettato le popolazioni indigene, rendendole di fatto schiave e macchiandosi di gravi episodi di violazione dei diritti umani. Si tratta di un dibattito che interessa anche altri Stati del Continente americano. Voglio però ricordare che, negli anni Trenta, a proporre l'abolizione del Columbus day fu il Ku klux klan, in odio alla popolazione italiana immigrata. Tale dibattito si è elevato a livello nazionale, in particolare in queste ultime settimane, intrecciandosi con episodi di vandalismo nei confronti di statue dedicate a Colombo in diverse località degli Stati Uniti e legandosi a pagine ancora controverse della storia americana, su cui periodicamente si accende un un serrato dibattito. Anche in Argentina, qualche anno fa, ci fu una polemica simile, e la statua di Colombo, che era davanti alla Casa Rosada, fu effettivamente spostata e, al suo posto, è stata messa la statua di una *leader* indigena. Alcune municipalità sono giunte in questi anni alla decisione di sostituire le celebrazioni del Columbus day, oggetto ogni anno di una *proclamation* presidenziale, con la Giornata delle popolazioni indigene. A Los Angeles, tuttavia, grazie all'impegno delle locali associazioni italoamericane, il Consiglio municipale ha istituito una Giornata dell'eredità culturale italoamericana, che verrà celebrata ogni anno presso quel Municipio, sempre il 12 ottobre. A fronte di questi avvenimenti, si registra una forte mobilitazione delle locali associazioni di italoamericani, come l'Order of sons of Italy o la National italian american foundation, così come la viva attenzione da parte dei rappresentanti eletti della collettività italiana residenti negli Stati Uniti, all'estero (CGIE) e dei Comites. Nel contesto di un quadro politico interno americano, caratterizzato da posizioni eterogenee sul tema della memoria di Colombo, si inserisce la presa di posizione molto chiara e netta del Presidente degli Stati Uniti, espressa attraverso l'atto di proclamazione della festività, pubblicato venerdì scorso. ha infatti voluto, da un lato, onorare la figura storica di Cristoforo Colombo e l'importanza delle sue imprese, sottolineando il coraggio e l'ambizione dell'esploratore, nonché l'impatto che la sua opera ha avuto per il corso della storia e per lo sviluppo degli Stati Uniti d'America. Allo stesso tempo, però, il Presidente ha voluto mettere al centro del proprio messaggio i sentimenti di stima, apprezzamento e amicizia nei confronti dell'Italia, patria di Colombo, definita definita «forte alleato e valoroso *partner* nella promozione della pace e della prosperità nel mondo». Infine Trump ha ricordato il contributo vitale apportato dalla comunità italoamericana alla cultura, allo sviluppo economico e alla società degli Stati Uniti. Nella giornata di ieri le manifestazioni si sono svolte regolarmente nelle principali città americane, senza registrare significative manifestazioni di protesta. A New York, in particolare, la presenza del sindaco de Blasio e del governatore Cuomo, accanto all'Ambasciatore d'Italia, testimoniano il rispetto per la memoria storica di Colombo e l'amicizia e la vicinanza delle istituzioni americane nei confronti del nostro Paese. Pur riconoscendo il carattere esclusivamente interno agli Stati Uniti della vicenda legata al mantenimento o no del Columbus day presso alcune municipalità statunitensi, la Farnesina ha costantemente seguito con grande attenzione la questione, come fece quando

Lo stesso ministro Alfano, che ha espresso nei giorni scorsi il proprio apprezzamento per le parole del presidente Trump, era già in precedenza intervenuto a proposito degli atti di vandalismo a danno delle statue di Colombo, sottolineando il carattere storico e simbolico dell'esploratore italiano. Venerdì 22 settembre, in occasione della sua presenza a New York per i lavori dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, si era infatti recato personalmente a rendere omaggio a Cristoforo Colombo a Columbus Circle, nel cuore di Manhattan, di fronte all'ingresso del Central Park,

La figura e l'impresa di Cristoforo Colombo sono state anche ripetutamente richiamate dall'ambasciatore italiano Armando Varricchio in occasione di diversi interventi pubblici come, ad esempio, durante il ricevimento ospitato dal sindaco di New York in occasione della giornata del patrimonio culturale italiano ovvero in occasioni più riservate e, da ultimo, nel ricevimento organizzato per la celebrazione dell'identità italoamericana (nei giorni che hanno preceduto la proclamazione ufficiale del Columbus day da parte di Donald Trump), alla presenza di numerosi membri del Congresso americano, di alti funzionari della Casa Bianca e consiglieri del Presidente e delle principali L'ambasciatore ha in tali occasioni sottolineato come americani, italiani e italoamericani debbano tutti sentirsi orgogliosi per lo straordinario contributo fornito da Cristoforo Colombo, che con la sua spedizione ha unito sponde fino ad allora separate, favorendo lo scambio di idee e culture. L'impegno comune delle istituzioni italiane e delle associazioni di italoamericani è quindi quello di sensibilizzare, nei modi e secondo le circostanze più appropriate, sia le istanze di Governo che la società civile statunitense sul profondo significato che in tutto il Paese le comunità italoamericane attribuiscono al Columbus day, quale giorno di riconoscimento del contributo degli immigrati italiani allo sviluppo degli Stati Uniti e dell'amicizia tra i nostri due popoli. Inoltre, come ha scritto ieri Gianni Riotta su «La Stampa», la storia non può diventare - io credo - una clava per la cronaca. Cristoforo Colombo non può essere giudicato con criteri attuali: era figlio del suo tempo. Sappiamo tutti cosa accadde in quella che è oggi l'America del Nord e l'America latina: schiavitù, massacri, dispersione degli amerindi, soprattutto morte dovuta al contagio con le nostre malattie. È il portato della colonizzazione europea, che ha una sua storia che resta una realtà con cui fare i conti, ma non si esorcizza abbattendo statue. In un'epoca di ossessioni identitarie, tutto viene riutilizzato e manipolato, anche la storia del passato, in nome di battaglie culturali o ideologiche odierne. La storia va letta e discussa nel contesto in cui si svolse e non riletta e revisionata a scopi politici o ideologici. Questo lo fanno i totalitarismi, come il fascismo che rinverdì il mito di Roma imperiale per giustificare la propria politica lo fanno i fondamentalisti odierni che rileggono le pagine dei libri sacri in maniera letteralistica per giustificare le proprie nefandezze e sognano una mitica età dell'oro che che oggi diviene incubo e che, tra l'altro, non è mai esistita. La storia è sempre contraddittoria, legata alla vita e non può essere essenzializzata, cioè congelata a elementi immutabili. Cristoforo Colombo fece un viaggio che nessuno voleva o sapeva fare e sbarcò su terre dove vivevano milioni di nativi che avevano la loro storia e la loro cultura. L'incontro - lo sappiamo - non fu felice all'inizio e per secoli ci furono rapine e saccheggi, ma da lì è nata l'attuale America, un mosaico di popoli che, alla fine, si sono mescolati e hanno rielaborato la loro cultura. Si tratta di Paesi diversi, se guardarti da vicino.

ma non storicizzati. Non si tratta di giustificare, ma di ricollocare. Colombo è il simbolo delle nostre collettività all'estero, molto più sentito - dobbiamo dirlo all'estero che in Patria. Anzi, in Europa ancora si discute se fosse italiano o spagnolo. Per gli italoamericani rappresenta il precursore, il primo tra loro a sbarcare su quelle coste, ma loro non pensano come lui. Come tutti gli americani di oggi, sono sensibili ai diritti delle minoranze, e anche gli italoamericani subirono gli effetti di un incontro gli effetti di un incontro difficile con gli Stati Uniti della loro epoca. Oggi sono riconosciuti come una parte importante della comunità degli Stati Uniti, ma l'inizio - lo sappiamo - fu difficile: niente di paragonabile con ciò che accade agli amerindi, ma comunque difficile. È questo il portato di ogni mescolanza, scontro e incontro assieme. Oggi siamo tutti più coscienti del fatto che occorre rispettare tutti e stimare la cultura di tutti, più incontro che scontro, ma la storia non si cancella buttando giù statue e ricordi. C'è stata un'epoca in cui gli europei credevano di essere superiori a tutti gli esseri umani; oggi non più. C'è stato un tempo in cui pensavano che la schiavitù fosse giusta; oggi non più. È il frutto di quell'incontro durato secoli e millenni. Tra le sofferenze si costruisce l'unità emotiva e giuridica dell'essere umano. La storia non è tema da tribunali, ma di coscienza comune sempre in divenire. *(Applausi

Signora Presidente, la ringrazio per l'appello che ha rivolto all'Assemblea, nel quale il nostro Gruppo si riconosce pienamente. Cercherò, quindi, di essere estremamente sintetico.

condiviso molti degli argomenti che le altre mozioni hanno portato all'attenzione dell'Assemblea sono state tutte ampiamente riprese nell'intervento del rappresentante del Governo. Da un punto di vista politico, credo che il rappresentante del Governo abbia fatto bene a riprendere le considerazioni del Presidente degli Stati Uniti d'America della scorsa settimana e ancor meglio ha fatto a richiamare quei valori di libertà storiografica che sono valori irrinunciabili della concezione liberale, democratica e civile della storiografia. Cristoforo Colombo appartiene certamente - è uno dei simboli più alti - alla nostra identità nazionale. Un'identità che non è così angusta, così meschina e così strumentale da essere sacrificata o sacrificabile a esigenze di correttezza politica o di inseguimento di questo o quel terzomondismo. La libertà storiografica è una libertà di opinione irrinunciabile, e proprio in nome di essa, insieme all'amico Carlo Giovanardi, ci ha fatto piacere che l'Assemblea del Senato potesse avere all'ordine del giorno l'esame di questi atti in

riprovazione per quanto avvenuto negli ultimi tempi negli Stati Uniti, dove centinaia di statue raffiguranti Cristoforo Colombo hanno subìto danneggiamenti e si è avuta notizia che numerose amministrazioni cittadine ne hanno chiesto la rimozione.

accusato di essere la causa e il simbolo delle persecuzioni subite dai nativi indigeni nei secoli successivi. Allo stesso modo, mi sembra segno di singolare ottusità richiedere l'abolizione della festa del Columbus day, giornata di festa nazionale sin dal 1937, che rappresenta un momento di gioiosa celebrazione per la comunità italiana negli Stati Uniti. L'uso politico della storia si configura sempre come un abuso e queste figure devono essere consegnate alla ricerca libera e ai libri di storia. È quindi auspicabile che il Governo italiano attivi le sue rappresentanze diplomatiche e culturali, da un lato, per favorire la conoscenza storica di Colombo e, dall'altro, per salvaguardare la sua memoria, le statue e la festa come segno perpetuo dell'amicizia tra il popolo italiano e quello statunitense, dal momento che la sua figura rappresenta un tangibile patrimonio dell'umanità.

in atto negli Stati Uniti, ribadisco il giudizio negativo sulla storia fatta in casa per compiacere prima se stessi e poi certi circoli cittadini che, nel fomentare la polemica, in nome dei diritti dell'uomo finiscono per rasentare l'ostracismo della storia, il razzismo ideologico e il negazionismo. È recente e va stigmatizzata pure da parte nostra la presa di posizione della presidente della Camera Boldrini sulla necessità di abbattere l'edilizia di

le posizioni che possano vantare nel mondo accademico quelle che noi chiamiamo le pezze d'appoggio, le pezze documentali. Tutto questo è pratica accademica e credo che arrogarci il diritto di avere una verità in tasca

possibile grazie soprattutto al sostegno di un altro Stato che non era l'Italia e è quindi parte di una storia comune del Mediterraneo, europea e mondiale, come tutte le storie

Mi chiedo però come mai in quest'Aula si manifesti attenzione nei confronti delle nostre comunità italoamericane a seguito di fatti così eclatanti

sono stati operati tagli per le attività di diffusione della nostra lingua e della nostra cultura nel mondo. Questo problema, infatti, prima che essere un problema politico, politico, è culturale. È inutile che scriviamo mozioni in cui impegniamo politicamente il Governo ad attivarsi nel quadro della normativa vigente negli Stati Uniti: Uniti: è un discorso di promozione della nostra lingua e della nostra cultura e, quindi, di sostegno alle nostre comunità italoamericane attraverso la rete delle ambasciate, dei consolati e degli istituti di cultura, che sono fondamentali per per far sì che non si arrivi a questo punto. Mi chiedo allora come mai non ci si sia indignati e come mai il vice ministro Giro non abbia fatto sentire forte e potente la sua voce quando sono stati operati questi tagli.

che chiede proprio che siano assegnate risorse finanziarie e umane, anche attraverso una riorganizzazione delle funzioni all'interno dei nostri consolati e delle nostre ambasciate, degli istituti di cultura, delle nostre scuole di italiani all'estero, dei nostri dipartimenti nelle università

fenomeni. Io sono molto d'accordo con il Sottosegretario quando dice che la storia non si riscrive abbattendo le statue. Ma non la si riscrive e certe cause non si perorano neanche

i nativi americani come «penne rosse» non porta proprio l'acqua al nostro mulino, perché in questa accezione ci vedo tutta la dinamica colonialista e neocolonialista che ha voluto vedere in quelle persone delle comunità

sostenere le nostre comunità italoamericane, ma perché li troviamo di poca utilità. Fatta questa richiesta, il nostro voto, se si procederà per parti separate, sarà favorevole su alcuni punti e di astensione su altri.

di italiani residenti negli Stati Uniti d'America a seguito di tutta una serie di interventi negativi sulla memoria di Cristoforo Colombo e non solo

nell'ottica di promuovere il progresso dell'umanità, abbiamo rilevato con grande preoccupazione culturale il fatto che ci potesse essere un revisionismo storico orientato forse più

Siamo soddisfatti che il Parlamento recepisca un'istanza che abbiamo immediatamente sollevato anche sulla spinta di larghissima parte dell'opinione pubblica attraverso numerosi articoli di stampa.

tra la comunità italiana e la storia degli Stati Uniti d'America e di altre Nazioni americane assolutamente positivo, ricordandone l'apporto importante dato alla loro economia, alla cultura

l'immagine della straordinaria unione sempre esistita tra i sentimenti italiani e i sentimenti del popolo nordamericano.

naturalmente pacifiche e assolutamente civili, dinanzi alla Casa municipale di New York e in altri luoghi importanti degli degli Stati Uniti d'America. Confermiamo, quindi, l'adesione all'ordine del giorno unitario, che consideriamo opportuno anche nei tempi - come lei, Presidente, ha sottolineato - perché viene approvato tempestivamente prima della ricorrenza del 12 ottobre, nonché importante per l'italianità, che deve essere difesa sempre e in ogni caso. L'italianità è la storia d'Italia, anche dentro le mura di casa nostra, perché qualcuno vorrebbe, ancora una volta, rivedere la storia del nostro Paese in chiave di strumentalizzazione politica. I monumenti della storia non possono essere soggetti alle bizze della cronaca. Quella è storia, mentre quella di oggi, quella che noi scriviamo è cronaca, sperando di poter far sì che un domani diventi, essa stessa, storia.

oggi l'attenzione al «politicamente corretto» fa salire sul banco degli imputati perfino Cristoforo Colombo, lo scopritore del Nuovo Continente; un padre fondatore e statista come Benjamin Franklin e George Washington, al quale è dedicata addirittura la capitale federale, l'amatissimo sindaco di New York, l'italoamericano Fiorello La Guardia, il cui nome è stato dato all'aeroporto principale della Città. Colombo, a lungo venerato, oggi è considerato un colonizzatore imperialista, che ha sterminato senza pietà le popolazioni autoctone monumenti a Franklin e Washington sono da demolire perché essi erano proprietari di schiavi, cosa che oggi farebbe inorridire, ma che all'epoca era considerata normale. Oppure abbattiamo anche le statue di Giulio Cesare, grande condottiero, ma anche sterminatore dei Galli. È sbagliato giudicare Colombo con i principi odierni, essendo vissuto nel 1400 e, e, di fatto, la statua a lui dedicata ricorda agli italoamericani il loro contributo nel costruire New York e le altre città, ed è l'omaggio degli immigrati italiani alle città che hanno edificato per la loro parte. La comunità italoamericana fa scudo intorno a Colombo, considerandolo un proprio simbolo distintivo. Le associazioni italoamericane hanno già manifestato nelle diverse città, assicurando di essere pronte a combattere per evitare la rimozione dei monumenti al navigatore genovese. Tra l'altro, nelle celebrazioni del Columbus day, hanno anche incassato il sostegno di Trump e si sono elevate in una corale, accorata, potente difesa. Hanno ricordato - come ha detto bene il Vice Ministro - come decenni fa fosse proprio il Ku Klux Klan a protestare contro Colombo, simbolo degli italiani, considerati etnia inferiore. inferiore. Noi italiani, che la Patria non l'abbiamo lontana, dovremmo imparare da loro a difendere la nostra storia. E bene facciamo oggi in quest'Aula a discutere le mozioni Quando gli uomini, con i propri simboli, sono consegnati ai libri c'è poco da rimuovere: perderemmo un pezzo di storia. C'è solo da studiare e capire e le tracce, anche fisiche, possono aiutare. La storia e i monumenti ricordano alle nuove generazioni i contributi che i nostri avi hanno dato e la storia ci insegna il passato, a come affrontare il futuro e, in altri termini, a non ripetere gli errori del passato. Lasciamo le statue alla storia. La politica pensi al futuro. Per questi motivi, il Gruppo del Partito Democratico esprimerà voto favorevole all'ordine del giorno condiviso, concordando pienamente sulle premesse e sul dispositivo.

Ricordo un discorso sentito così, di sera, tra mamma e papà, un discorso fatto quando noi bambini - eravamo in cinque - non eravamo presenti. Ricordo quella sera che la mamma diceva al papà: "Non sarebbe meglio mandare i bambini a Belluno?" Mi sono fermata a origliare. Perché la mamma voleva mandarci via? Cosa avevamo fatto? La voce di papà rispose: "Cosa vuoi che mi importi? Se cade la diga, parte anche Belluno; se dobbiamo morire, meglio farlo tutti insieme". Era un discorso troppo duro e forte, almeno per me, incomprensibile. Guardavo la diga e pensavo: "Come può farci del male e farci morire?"». Queste, Presidente, sono le parole di Micaela, una bambina sopravvissuta al disastro del Vajont. Presidente, onorevole Vice Ministro, colleghe e colleghi, mi rivolgo a tutti e chiedo all'Aula di unirsi al ricordo, doveroso per noi che rappresentiamo le istituzioni, del 54° anniversario dalla catastrofe del Vajont, celebrato ieri nei luoghi del ricordo con la deposizione delle corone e la messa solenne al Sacrario monumentale delle vittime del Vajont. È stato celebrato ieri nel silenzio del dolore che ancora accompagna i pochi superstiti in vita e tutti coloro che in quei luoghi hanno continuato a vivere dopo la tragedia del 9 ottobre del 1963: 1.910 morti, una generazione spazzata via, paesi cancellati dalla furia di un'onda che ha superato la diga portando con se solo morte e disperazione; nessun risarcimento ai sopravvissuti. Quella diga, Presidente, è ancora lì, integra, ma la montagna si è ribellata all'avidità di uomini consapevoli di ciò che stava accadendo, e non certo all'incuria. Presidente, ho chiesto il rispetto delle vittime sepolte nel Cimitero monumentale attraverso un contributo che aiuti i volontari nella cura e manutenzione di quel luogo sacro.

Lei, però, è anche lo stesso uomo che si è abbandonato a facili polemiche, soprattutto su Twitter, e non solo con persone del calibro di Saviano, ma anche con un cantante, con artisti, politici e persino un minorenne.

Segue forse la strategia del «nel bene o nel male, basta che se ne parli»? Non le dà alcun fastidio che i toni delle comunicazioni politiche si siano tanto abbassati? Oggi assistiamo a un teatrino piuttosto malmesso con cariche istituzionali che usano turpiloquio

è che ogni volta che un politico parla e scrive, in quel momento giustifica il pensiero di quei milioni di italiani che pensano che siamo una manica di incompetenti, strapagati e viziati, o meglio "vitaliziati". Se noi parliamo e agiamo come tutti, se non offriamo niente di meglio di chiunque altro e non mostriamo un po' di dignità, competenza e dedizione, allora perché guadagniamo Non potremmo allora moderare un pochino i toni? Lo scambio di idee deve essere per forza così becero? E parlo non dello specifico evento che ho prima

Sui giudizi sulla mia competenza gli elettori da decenni si esprimono in maniera più generosa di quanto scoprirà tra qualche settimana la senatrice Bencini nei suoi confronti. Ci avviamo infatti alle elezioni e io le faccio i migliori auguri, ma vedo il suo percorso accidentato e difficile. Per quanto riguarda la vicenda cui si fa riferimento, ci sarà una contesa in sede giudiziaria per decidere se la parola «pregiudicato» si può applicare solo a condanne penali - come alcuni ritengono, ma la legge non afferma - o anche a condanne definitive in sede civile. Lo scrittore in oggetto, Saviano, ha avuto una condanna definitiva per un plagio di alcuni articoli in un

farci incardinare in sede parlamentare, benché a fine seduta, questa *querelle*. Saviano ha detto letteralmente, senza essere interrotto dal conduttore, che coloro che sono contro lo *ius soli*, della Lega e non solo - io faccio parte del «non solo», perché non sono della Lega - sono dei teppisti. Non so se questo sia un linguaggio - lo dico in presenza del senatore Zavoli - da prima rete nei confronti dei partiti, con il massimo ascolto la domenica sera. Inoltre devo anche ringraziare Saviano, perché diventerò ricco e devolverò i proventi delle cause agli orfani dei Carabinieri. Dopo il suo *post* su Facebook, infatti, ho ricevuto circa 3.000-4.000 insulti pesantissimi («ti ammazzeremo, ti impiccheremo, ti spareremo»), con nomi e cognomi, perché scrivono a Saviano pensando che io non legga. Io ho mandato anche al presidente del Senato Grasso e alla presidente della Camera Boldrini (che giustamente fa le campagne antiodio)

e quelli che continueranno a insultare saranno denunciati uno per uno. Assocerò gli insulti che sto ricevendo alle iniziative della presidente Boldrini, che condivido, sulle campagne d'odio. Io ho detto un fatto di una sentenza, mentre gli altri alimentano campagne d'odio. La senatrice Bencini - come dire - la sventurata parlò,

Signora Presidente, nel 2013 il Ministero dell'interno ha individuato il Comune di San Giuliano di Puglia in Molise come sede di un centro di accoglienza per i richiedenti asilo, con una disponibilità ad accogliere da 500 a 1.200 persone. A tale scopo, è stata bandita una gara per la ristrutturazione del villaggio in legno che, nel 2002, ospitò gli sfollati dopo il terribile terremoto che costò la vita a 27 bambini e a una maestra. Io ho presentato diverse interrogazioni nelle quali ha fatto presente l'impraticabilità di una simile iniziativa, che andrebbe a collocarsi in un Comune di appena 800 abitanti, in un territorio sismico, privo di adeguati presidi sanitari e di ordine pubblico e socialmente inidoneo ad accogliere un numero così elevato di richiedenti asilo. Negli ultimi tempi si sono moltiplicate le manifestazioni contro questo progetto e tre Comuni limitrofi hanno deliberato la loro contrarietà. È di ieri la dichiarazione del ministro dell'interno Minniti secondo la quale, vista la drastica riduzione degli sbarchi di migranti sulle coste del nostro Paese - si parla del 90 per cento - il suo obiettivo è quello di chiudere i centri di accoglienza per migranti, per passare all'accoglienza diffusa sul territorio.

del 5 aprile 2017 e che vengano fermate le procedure per la costruzione del centro di accoglienza a San Giuliano di Puglia.